onorevoli senatori, anzitutto ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito che ha posto. Passo quindi a illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente proprio i criteri di computo dell'assegno unico universale nell'indicatore

Infatti, l'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, in combinato disposto con la previsione del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, dispone, tra l'altro, che i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e quindi esenti, per ragioni diverse dalle condizioni di disabilità, rientrino nel calcolo dell'indicatore della situazione reddituale dell'ISEE.

per tutte le altre prestazioni, proprio perché il decreto legislativo di varo dell'assegno unico universale non ha al suo interno una previsione che dà risposta a questa criticità.

l'istituto, in quanto ente erogatore, è tenuto a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della stessa prestazione percepito nel secondo anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) rapportato al corrispondente parametro della scala equivalente. La norma dispone infatti che gli enti erogatori

delle mensilità dell'assegno unico universale, per l'anno 2024 l'ISEE non terrà conto di quanto ricevuto per lo stesso assegno nel costo dell'anno 2022. Voglio sottolineare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segue con estrema attenzione e monitora l'efficacia degli strumenti di sostegno messi in campo a favore delle famiglie. Siamo anche consapevoli che questa è una prima risposta immediata per non avere una ricaduta

natalità. Le leggi di bilancio che si sono succedute negli ultimi due anni, grazie all'impegno di tutto l'Esecutivo, hanno ampliato la fruibilità dell'assegno, in particolare per le famiglie numerose, per quelle con un figlio disabile e, in determinati casi, anche per le famiglie con figli al di sotto dei tre anni.

gli sforzi sono tanti, ma non crediamo che siano ancora sufficienti a poter riconoscere ad ogni famiglia il diritto di procreare e mettere al mondo bambini, quindi l'impegno del Governo sarà continuativo per tutta la legislatura, per dare maggiore sostanza e opportunità a ciascun cittadino.

È dunque intenzione del Governo lavorare in sinergia per individuare le aree di intervento critiche e prospettare contestualmente possibili soluzioni. Sappiamo che qualsiasi azione che abbia come oggetto l'ISEE dev'essere particolarmente studiata e attenzionata sia nel superamento delle criticità attualmente esistenti, sia nell'impatto e nelle ricadute che evidentemente si ripercuotono sui diversi provvedimenti e le diverse prestazioni che vedono in gioco l'ISEE: abbiamo visto come viene utilizzato per moltissimi interventi e moltissime riforme

È diventata una misura equa, perché prima i figli dei lavoratori autonomi non ricevevano sostegni adeguati alla loro

sta funzionando molto bene. Dopo il primo anno di attuazione abbiamo avuto risparmi; durante il Governo Draghi quei risparmi non erano stati utilizzati, mentre voi avete utilizzato circa 600 milioni

Nessun'altra misura è così efficace nella lotta alla povertà come quella che abbiamo messo in campo, a dimostrazione che non bisogna fare riforme *spot*, ma strutturali, che durino nel tempo, che sostengano i cittadini per tutto l'arco della loro vita. C'era un problema in sospeso, tra gli altri, che non

e con l'altra prende.

semplicemente, com'era scritto nella delega, che ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, il computo dell'assegno debba essere differenziato nell'ambito dell'ISEE, fino all'azzeramento. Era scritto così nella delega,

Signor Presidente, ringrazio l'onorevole interrogante che, ponendo una questione relativa al tribunale di Vicenza, in verità ne pone una più complessiva in ordine alla scopertura del personale amministrativo e delle delle piante organiche dei tribunali d'Italia, in merito evidentemente anche all'impatto che può avere sull'abbattimento dell'arretrato e al *disposition time* in relazione al PNRR. Ringrazio l'onorevole interrogante perché consente al Governo di rappresentare l'imponente lavoro di reclutamento, in particolare del personale amministrativo,

di imponente attività di reclutamento avviata dal Ministero della giustizia, considerato che sono state effettuate 10.248 assunzioni di risorse umane nell'intero territorio ma è una quantificazione che può definirsi per difetto e non certamente per eccesso, perché a queste vanno aggiunte le assunzioni concernenti gli addetti all'ufficio del processo e il personale a supporto dell'ufficio del processo, che sappiamo essere stato immaginato proprio per affrontare l'abbattimento l'abbattimento dell'arretrato e quindi, a fronte delle 10.248 assunzioni relative al personale più propriamente detto amministrativo, devono essere aggiunte le 12.354 unità relative ai profili di addetto per l'ufficio del processo e di

contrastare il fenomeno dell'arretrato. Venendo *in* *medias res* e più puntualmente alle risposte dovute in ordine al tribunale di Vicenza, va ricordato che a fronte di una dotazione organica di 142 unità, attualmente prestano servizio 90 risorse umane. Nel computo complessivo delle risorse impiegate nel tribunale di Vicenza, non vengono però computate le ulteriori 48 unità assunte a tempo determinato nell'ambito dei reclutamenti degli addetti all'ufficio del processo (34 unità) e del personale a supporto dell'ufficio del processo (14 unità). Le vacanze registrate nei vari profili interessano poi le seguenti figure professionali: ausiliari, otto vacanze su 16 posti in organico; assistente giudiziario, 17 vacanze su 47 posti in organico; cancelliere, 17 vacanze su 22 22 posti in organico; funzionario giudiziario, sette vacanze su 31 posti in organico. Fortunatamente, invece, le figure professionali del direttore, dell'operatore giudiziario e del conducente di automezzi risultano soddisfatte. In data 26 luglio 2023 è stato pubblicato un interpello nazionale per 9.739 posti vacanti rivolti al personale dell'organizzazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sindacale del 15 luglio 2020. Per la Regione Veneto nel suo complesso sono stati resi disponibili 474 posti e per il tribunale di Vicenza sono stati pubblicati 35 posti, segnatamente sette di assistente giudiziario, 17 di cancelliere, sette di ausiliario e quattro di funzionario giudiziario, che purtroppo non sono stati oggetto di scelta da parte dei dipendenti. Peraltro, nell'ambito della procedura di interpello, si sono concretizzati trasferimenti in uscita di quattro unità di personale dall'ufficio in esame presso altri uffici giudiziari, uno ausiliario e tre assistenti giudiziari. Si rimarca, in ogni caso, che dal piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 emerge chiaramente - inequivocabilmente, direi - la volontà di questo Dicastero di sopperire quanto più possibile alle carenze di personale amministrativo e ciò di certo determinerà effetti positivi a ricaduta anche sugli uffici giudiziari di Vicenza. In questa direzione va certamente la previsione di procedure volte alla stabilizzazione del personale amministrativo assunto

Le attività di reclutamento previste nell'arco temporale dal 2023 al 2025 riguardano complessivamente 1.051 unità nell'area dei funzionari, 6.624 nell'area degli assistenti, 179 nell'area dei dirigenti, per un totale di 7.854 risorse umane. A ciò è da aggiungere il contingente di 3.691 unità di personale amministrativo non dirigenziale, per le quali l'autorizzazione a bandire e ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali è prevista da varie fonti normative divise in 1.967 funzionari e 1.724 assistenti. Si segnala poi che in data 28 febbraio 2023 è stata disposta la proroga della scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal personale assunto con la qualifica di operatore giudiziario e la contestuale assunzione

per pensionamento di personale, ovvero per altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (dalla maternità alla malattia), l'organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari in difficoltà potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale prevista dall'articolo 20

collaborazione - che cito testualmente - in tema di selezione e di reclutamento di personale, attraverso il possibile perfezionamento di procedure concorsuali uniche per i reciproci coincidenti fabbisogni in termini di inquadramento e profilo professionale della Regione Veneto, degli uffici giudiziari operanti nel Veneto e/o il convenzionamento per l'utilizzo reciproco delle graduatorie in relazione ai concorsi direttamente espletati da ciascuna delle parti parti firmatarie. Lo scorrimento di graduatorie regionali dovrebbe garantire un successo maggiore rispetto all'interpello di cui parlavo prima, che purtroppo non ha dato esito positivo, non certamente per cattiva volontà del Ministero, ma perché sono state scelte altre sedi. In forza della convenzione del 30 giugno 2023,

di 30 posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria B, posizione economica B3. Nelle giornate dal 5 al 13 luglio 2023, gli idonei interessati a entrare nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di assistente giudiziario hanno partecipato alla procedura di scelta tra i 69 posti messi a disposizione dall'amministrazione giudiziaria del distretto della corte d'appello di Venezia, di cui tre individuati presso il tribunale di Vicenza. Si rappresenta che, all'atto della presa di possesso, avvenuta il 12 settembre 2023, purtroppo, una sola delle tre unità contemplate ha sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro. Sempre nel solco dell'accordo richiamato con la Regione Veneto, è prevista la facoltà di attingere dalle graduatorie regionali in corso di validità per l'assunzione di 28 conducenti di automezzi nell'intero distretto. Peraltro, sono in atto le opportune interlocuzioni per l'ulteriore utilizzo della graduatoria regionale, al fine di assumere ulteriori unità nel profilo di assistente giudiziario. Si evidenzia altresì che, in virtù dello scorrimento per 743 unità

otto unità presenti nella graduatoria del distretto di Venezia. La presa di servizio degli aventi diritto è avvenuta il 12 marzo 2024.

interrogazioni sugli organici di magistrati e personale amministrativo del tribunale di Vicenza, ottengo la relativa risposta e bene o male tutte le volte in questi anni è stato garantito impegno. Sono

media del 27,63 per cento. Le do quella attuale, a ieri, così come mi è stata confermata dai capi degli uffici giudiziari vicentini. Partiamo dal tribunale: i dipendenti a tempo indeterminato effettivi presenti sono 77 su 142, quindi con una scopertura del 45,7 per cento, pressoché doppia rispetto alla media nazionale. Tra l'altro, alcuni di questi, che sono a tempo determinato, hanno vinto il concorso all'Agenzia delle entrate, dove passeranno a breve, quindi questa scopertura si accentuerà. Le do anche i numeri della procura: allo stato, la scopertura del personale amministrativo è pari al 38,89 per cento (anche questa è superiore alla media nazionale); sono 54 i posti previsti, 21 quelli vacanti le unità in posizione di distacco presso altri uffici. La situazione è quindi drammatica. Parlo del personale amministrativo, che oggi, per certi versi, soprattutto nelle realtà del Nord

per cercare di ridurre l'arretrato e conseguire gli obiettivi concordati con l'Europa e con il PNRR falliscono. Questo consente anche una riflessione più generale a noi che ci occupiamo di giustizia e cerchiamo di dare il nostro meglio nella legislazione: forse molti - anzi, anzi, sicuramente la gran parte - dei problemi della giustizia sui temi dello smaltimento e dell'arretrato possono essere affrontati meglio con una migliore organizzazione del personale sul territorio,

più che un impegno ad aprire tribunalini, magari diffusi sul territorio, divisi fra tre o quattro sedi locali, distanti centinaia di metri lineari l'una dall'altra, l'impegno del Governo dovrebbe andare proprio su questi temi concreti. *(Applausi)*.

Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti che mi danno modo di chiarire ciò che credo sia frutto di un *misunderstanding*. Gli onorevoli interroganti lamentano il mancato scorrimento di una graduatoria

era impossibile, perché avremmo violato il dettato legislativo. Dev'essere infatti sottolineato che l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è regolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 146 del 2000 ed avviene

al quale cioè può partecipare solo chi è già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il decreto del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 1° ottobre definisce poi le procedure e le modalità di svolgimento sia dei concorsi pubblici sia dei concorsi interni, con riferimento

Con riguardo quindi alle procedure di selezione indicate nell'atto di sindacato ispettivo, segnalo che il concorso per 120 allievi di commissari di Polizia penitenziaria è stato bandito per la copertura dei posti da assegnare mediante concorso pubblico nel limite massimo del 70 per cento della pianta organica, poi aumentati a 132 rispetto ai 120 iniziali, avvalendosi dell'ulteriore facoltà di aumentare del 10 per cento. I vincitori del concorso pubblico sono stati avviati al corso di formazione; mediante scorrimento della graduatoria, come effettivamente indicato, si è proceduto alla sostituzione dei candidati

interno della graduatoria, ma, arrivati al limite del 70 per cento, siamo stati costretti dal dettato legislativo ad aprire un'altra procedura interna per titoli e anzianità relativa invece alla quota del 30 per cento per l'assunzione dei funzionari.

gli aspetti procedurali e normativi che hanno giustificato l'indizione di un concorso successivo al primo.

quella degli organici della Polizia penitenziaria, soprattutto in un momento come questo, in cui la situazione carceraria italiana è in gravissima sofferenza. Sappiamo quanto sono importanti questi concorsi.

che comporta un incremento costante e continuo dei detenuti nei penitenziari italiani. Purtroppo infatti questa è la situazione che stiamo registrando. anche alle condizioni di lavoro dei nostri agenti di Polizia penitenziaria, che fanno un lavoro encomiabile e che ringraziamo per il servizio che svolgono nei nostri penitenziari. È un lavoro che si svolge in condizioni sempre più difficili e drammatiche, non solo per la carenza di personale, ma soprattutto per le condizioni in cui versano i nostri penitenziari e per l'aumento dei detenuti,

di politica criminale di questo Paese. Infatti, se non intraprenderemo un percorso diverso, che porti non dico a una riduzione, ma quanto meno a una stabilizzazione del numero complessivo di detenuti,

- Premesso che: da anni la situazione occupazionale delle professioni sanitarie, principalmente ospedaliere, riflette decenni di errata programmazione, in tema di reclutamento delle professionalità nel mondo della salute pubblica; il fenomeno dell'abbandono degli ospedali

qualificate, circa 80.000 professionisti mancano all'appello. Il calo del numero dei medici e il forte incremento di prestazioni da erogare, per effetto dell'aumento dell'aspettativa di vita e della cronicizzazione di tantissime patologie, in tutte le aree di specializzazione il mercato dei cosiddetti medici a gettone. Si definiscono gettonisti i medici che prestano la propria opera tramite cooperative contrattualizzate dalle strutture sanitarie pubbliche che vengono remunerati in proporzione alle singole prestazioni per la copertura dei servizi sanitari. È questo un sistema che, come così come è organizzato, non garantisce ai cittadini una buona qualità delle cure somministrate, visto che i medici vengono spesso utilizzati in servizi senza avere le necessarie competenze e non si prevede il rispetto dei riposi indicati dalla normativa europea. Tale pratica del gettonismo, particolarmente rilevante nel campo dell'emergenza urgenza, ha generato un perverso sistema che non permette ai servizi sanitari regionali di offrire un servizio di qualità in tempi accettabili. Signor Ministro, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ella ha significativamente aumentato i posti nelle università italiane per lo studio della medicina, continuando il *trend* intrapreso con gravissimo ritardo dai precedenti Governi, solo dopo la pandemia da Covid-19. Le borse per le specializzazioni mediche, in talune discipline, risultano superiori al numero dei partecipanti ai concorsi relativi e alcuni aggiustamenti intra specialità saranno necessari al fine del definitivo superamento del cosiddetto imbuto formativo, anche smettendo di pagare i medici tutti allo stesso modo.

(articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2023) volte, tra l'altro, a favorire la re-internalizzazione dei servizi sanitari, anche prevedendo delle premialità

Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti, che mi offrono l'opportunità di tornare su un tema che, come Ministro della salute e come medico, mi sta particolarmente a cuore, che è quello della valorizzazione delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale e del contrasto al fenomeno dei cosiddetti medici gettonisti. In merito a questo fenomeno, ricordo che, a seguito di attività ispettiva dei Nas, che ho disposto fin dal mio insediamento per contrastare l'abuso delle esternalizzazioni, con particolare riguardo all'affidamento a cooperative di interi reparti ospedalieri, specie nell'emergenza urgenza, su mio impulso questo Governo, con il decreto-legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023, ha per la prima volta dettato specifiche disposizioni volte a contrastare questo abuso. Come ricordava il senatore Zaffini, l'articolo 10 del decreto ha previsto la possibilità, per le aziende e gli enti del Sistema sanitario nazionale, di procedere alla esternalizzazione dei servizi stessi nei soli casi di necessità e urgenza, in un'unica occasione, senza possibilità di proroga laddove non sia possibile ovviare altrimenti alla carenza di personale sanitario. È inoltre prevista l'elaborazione, da parte del Ministero della salute con l'Anac, di apposite linee guida volte a ricondurre questi affidamenti entro limiti ben precisi. Inoltre questo Governo, nella consapevolezza di intervenire in maniera strutturale per reperire le risorse necessarie al sistema, per migliorare l'organizzazione dei servizi e far sì che il Sistema sanitario nazionale torni ad essere maggiormente attrattivo per i giovani, ha adottato, sin dal suo insediamento, diverse misure anche di tipo economico. Ricordo, a tal proposito, l'incremento della specifica indennità, con un impegno complessivo di 200 milioni di euro annui nella legge di bilancio 2024 per le particolari condizioni di lavoro presso i servizi di pronto soccorso. Ricordo, inoltre, l'estensione fino al 31 dicembre 2026 della facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico prevista per l'anno 2023, aumentate da 60 a 100 euro lordi, disponendo che tale incremento riguardi tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Per fronteggiare gli errori della programmazione del reclutamento del personale sanitario, reiterati per decenni, e il problema della carenza di medici, ho adottato specifiche misure volte a facilitare il reclutamento strutturale di medici del Sistema sanitario nazionale, riconoscendo la possibilità a coloro che hanno maturato un congruo periodo di esperienza presso i servizi di emergenza urgenza di partecipare ai concorsi. Inoltre, con il Ministro dell'Università, in intesa, abbiamo invertito il *trend* all'origine, incrementando gli accessi al corso di laurea in medicina e chirurgia e alle scuole di specializzazione, passando da 10.000 unità circa dell'anno 2019 alle oltre 18.000 di quest'anno accademico. Con riferimento, invece, al cosiddetto problema dell'imbuto formativo, delle specializzazioni mediche e del numero di borse di studio per l'accesso alle scuole di formazione specifica in medicina, oggi è del tutto superato grazie agli interventi posti in atto con la Missione 6 componente 2 del PNRR, che ha consentito il finanziamento di 4.200 contratti di formazione medico-specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con fondi ordinari e di 900 borse aggiuntive per la formazione specifica in medicina generale. Resta tuttavia ancora una criticità legata alla distribuzione dei contratti di specializzazione medica dovuti ad una minore attrattività di alcune specializzazioni rispetto soprattutto a quelle che offrono maggiori sbocchi lavorativi nel privato e nella libera professione. Mi si permetta di concludere che la prima frase del quesito postomi colpisce nel segno: siamo in questa situazione a causa di decenni di errata programmazione. Non c'è traccia, nelle manovre dell'ultimo decennio, di azioni concrete per aumentare i posti nella facoltà di medicina in vista del fisiologico *turnover*. Non c'è traccia di battaglie per l'abolizione dei tetti di spesa e nemmeno di generiche battaglie a tutela del Servizio sanitario nazionale, al netto di qualche *slogan*. La strada è quella che abbiamo tracciato fin dall'inizio. Il Sistema sanitario nazionale si sostiene con l'organizzazione, con la valorizzazione del personale e con la caccia alle inefficienze. Stupisce leggere che chi agita il fantasma di una crescente privatizzazione della sanità è proprio chi ha innescato la tendenza gettonistica, non facendo nulla per contrastare le esternalizzazioni e il proliferare di cooperative di medici a cottimo. il Ministro per la chiarezza della sua illustrazione. I medici non ci sono e ciò è dovuto a un difetto di programmazione. E non ci sono perché qualcuno ha stabilito che non si potessero sostituire quelli che andavano in pensione. E non ci sono perché, di punto in bianco, qualcuno ha deciso che quello che prima facevano tre, da un certo momento in poi lo potesse fare uno solo. Mancano i medici, ma mancano anche gli infermieri e gli operatori sociosanitari e questo è un problema che ci è stato consegnato. del vigore con il quale il Ministro sta affrontando il tema. Il ministro Bernini, da parte sua, ha provveduto ad aumentare molto i posti disponibili presso le facoltà di medicina. Ma il medico si forma in dieci anni, per cui i frutti di questo lavoro li vedremo, purtroppo, tra qualche anno.

È ovvio che alcune professioni - lo vediamo dal minor *appeal* dei corsi di specialità - siano meno appetibili; ebbene, quelle professioni, che sono veramente indispensabili però al Servizio sanitario nazionale - è inutile che le citiamo - andranno pagate di più. Dovranno essere pagati di più quei professionisti che hanno minore sbocco nell'attività privata, nella libera professione. So che di tutto questo il Ministro è perfettamente consapevole per il ruolo che svolge e gli garantisco la vicinanza del Parlamento e della mia Commissione per quanto di competenza, la necessità che su tali evidenti malfunzionamenti si intervenga con il vigore necessario. *(Applausi)*.

larghe fasce di popolazione su tutto il territorio nazionale, in quanto il problema sussiste da Nord a Sud. Va detto che il sistema delle prenotazioni *online* non funziona. I cittadini sono costretti a mettersi la mattina davanti al *computer* e a le ore 8,01 per cercare di prendere un agognato appuntamento, che il più delle volte non arriva; pertanto, i tentativi si susseguono di settimana in settimana. Ciò crea un clima di esasperazione e di rabbia, tant'è che, poi, molto spesso, soprattutto chi ha proprio necessità del passaporto è costretto

dell'interno*. Signora Presidente, la soluzione della questione dei tempi di rilascio dei passaporti è affidata all'attuazione del progetto Polis, citato peraltro dagli onorevoli interroganti, a cui il Governo ha dato avvio in questi giorni e che sarà progressivamente esteso a tutti i Comuni con meno di 15.000 abitanti ed in prospettiva anche a quelli con popolazione superiore su tutto il territorio nazionale. Grazie al progetto Polis i cittadini potranno richiedere o rinnovare il passaporto, presentando la documentazione direttamente agli sportelli di Poste Italiane, senza doversi recare in questura e con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio. L'attuale fase di sperimentazione, avviata in due Comuni in provincia di Bologna, ha già consentito il rilascio dei primi passaporti, anche con consegna al domicilio del richiedente. In attesa della piena attuazione del progetto Polis, prosegue il notevole sforzo organizzativo delle questure, accompagnato da ulteriori interventi di potenziamento delle risorse umane e strumentali a disposizione degli uffici. Come ricordato dall'onorevole interrogante, questo straordinario impegno è comprovato dal rilascio nel 2023 di 2.750.000 passaporti, cioè un milione in più rispetto a tutti gli anni del periodo pre-pandemico. I dati di quest'anno mostrano un *trend* in ulteriore miglioramento: sono stati emessi circa 250.000 passaporti al mese dall'inizio dell'anno, mentre nei primi dodici giorni di marzo ne sono stati emessi 113.000, con la previsione di chiudere il mese con oltre 300.000 documenti rilasciati. Aggiungo che, per venire incontro ai cittadini che hanno esigenze di un rilascio urgente (legato cioè a motivi di salute, studio, lavoro, turismo), è già operativa in 52 Province un'agenda *online* prioritaria. A partire dalla prossima settimana, le nuove modalità operative dedicate a tali esigenze saranno adottate su tutto il territorio nazionale e confidiamo in tal modo di realizzare una progressiva riduzione dei tempi di attesa. l'interrogante stesso ha sottolineato, si è reso necessario perché l'aumento esponenziale e ravvicinato del numero di istanze di rilascio di passaporti registrato - come ho detto - nel periodo postpandemico, ma anche a causa, ad esempio, di situazioni come la Brexit, ha fatto emergere la necessità di ridisegnare le procedure fino ad oggi utilizzate per snellirle, alleggerire le attività amministrative svolte dalle questure e renderle sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini. dato delle informazioni molto utili e decisive per quanto riguarda la soluzione di questo annoso problema. Il progetto Polis rappresenta sicuramente un grosso passo avanti.

una nuova opzione per la necessità del rilascio del passaporto per viaggi programmati entro trenta giorni, è sicuramente una soluzione molto utile, innovativa, che proprio in queste ore viene varata e che consentirà di risolvere almeno i problemi più urgenti. Fino ad oggi devo riconoscere che il personale delle questure - parlo per la mia città - è stato lodevole nell'impegno di di adempiere anche a richieste urgenti e questo ha consentito di tamponare almeno i casi più eclatanti. Certamente dobbiamo mettere a norma il sistema e consentire al cittadino, senza

con l'accusa di organizzazione e associazione con finalità di stampo terroristico. Naturalmente, approfitto per fare i complimenti, per l'intervento puntuale e preciso, al Ministero e alle Forze dell'ordine, che in più occasioni sono riusciti ad

A tal fine noi, come Gruppo Lega, abbiamo depositato un disegno di legge, l'Atto Senato n. 909, che di fatto mette in evidenza la possibilità di compiere quell'opera che nel nostro Paese è un po' complicata, nel senso che noi siamo sempre molto bravi ad intervenire nelle urgenze, ma nella prevenzione un po' meno: da una parte cercare di formare e preparare il personale docente in caso di situazioni di attacco e, dall'altra parte, indurre gli stessi studenti a comportamenti virtuosi in caso di emergenze. Questo non significa provocare allarmismi, ma significa semplicemente, come fanno altri Paesi, prepararsi in questa direzione. Il nostro è un progetto di legge, ma vogliamo capire - e per questo facciamo la domanda - se il Governo, il suo Ministero, intenda in qualche modo integrare un piano, che voi sulla prevenzione avete opportunamente studiato, anche sul fronte della preparazione e/o comunque dell'attenzione sugli istituti scolastici.

delle nostre Forze dell'ordine e testimonia la costante azione di monitoraggio e prevenzione realizzata sul fronte dell'estremismo e della radicalizzazione. Dopo il 7 ottobre - com'è stato ricordato - ho immediatamente disposto un rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo, riferiti agli obiettivi sensibili presenti sul territorio. E nella seduta del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato d'urgenza il 10 ottobre, con la partecipazione delle agenzie di *Intelligence*, sono stati approfonditi le possibili minacce e gli strumenti di prevenzione e contrasto. È stata effettuata una ricognizione degli obiettivi sensibili in Italia, che sono stati quantificati in oltre 28.000, 205 dei quali riconducibili ad Israele, in prevalenza sedi diplomatiche o centri religiosi. La minaccia terroristica, inoltre, è sempre oggetto di approfondimento nell'ambito del Comitato di analisi strategica antiterrorismo, anche in un quadro di collaborazione operativa con gli apparati antiterrorismo dei Paesi europei ed extra UE. La strategia di prevenzione messa in campo a più livelli non ha mancato di considerare il monitoraggio delle piazze digitali, dal quale emerge una preoccupante recrudescenza del sentimento anti-israeliano, una particolare attenzione rivolta anche ai possibili profili di rischio di infiltrazione terroristica nei flussi migratori. Sono state pertanto potenziate le attività interforze per i controlli delle frontiere marittime nelle principali aree di sbarco e negli *hot spot* nazionali, nonché delle frontiere terrestri, anche grazie al ripristino temporaneo dei controlli degli ingressi dalla Slovenia. L'impegno delle Forze dell'ordine è testimoniato dai risultati conseguiti dall'attività di contrasto, che dal 2023 a oggi ha portato all'arresto di 26 soggetti per terrorismo internazionale. La stessa attività di contrasto ha anche consentito, nel medesimo periodo, di eseguire provvedimenti finalizzati all'allontanamento dal territorio nazionale di 95 soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza, 45 dei quali proprio dal 7 ottobre scorso. Circa le pianificazioni di emergenza, lo scorso 18 settembre è stato approvato il nuovo piano nazionale di emergenza per la gestione di gravi turbative dell'ordine pubblico e di eventi di matrice terroristica. Alla pianificazione nazionale è seguita la rivisitazione dei piani di livello territoriale a cura delle autorità provinciali di pubblica sicurezza per la ricognizione di tutti gli obiettivi sensibili presenti nei singoli territori, per per verificarne il grado di esposizione a rischio, nonché per ogni altra possibile attività di prevenzione. È proprio in tale ultimo ambito che gli istituti scolastici potranno essere oggetto di indicazioni di dettaglio da parte delle stesse autorità provinciali.

*(PD-IDP)*. Signor Ministro, la città di Trieste costituisce un punto di arrivo della cosiddetta rotta balcanica, la quale interessa, ogni anno, molte migliaia di persone migranti: oltre 13.000 nel 2022 e 16.000 nel 2023, provenienti prevalentemente da Afghanistan, Subcontinente indiano, Regioni del persone che versano in condizioni tali da giustificare la condizione dello *status* di rifugiato. Un numero significativo di persone si ferma a Trieste e lì avvia il percorso di richiesta di protezione internazionale. Queste persone non accedono ad alcuna forma di prima accoglienza. Un numero elevato trova riparo in luoghi di fortuna fatiscenti, come il cosiddetto Silos, edificio diroccato che è divenuto insediamento informale. Le chiedo dunque, Ministro, sia a conoscenza del vero e proprio dramma umanitario che si sta consumando nel cosiddetto Silos di Trieste, quali siano le sue valutazioni al riguardo e se riconosca che finora nel Silos di Trieste si è consumato un dramma umanitario, con l'abbandono di molte persone che non hanno avuto - e al momento non hanno ancora - alcun tipo di assistenza dalle istituzioni, mentre gli unici aiuti vengono dal mondo del volontariato e delle associazioni laiche e religiose; se sia vero che l'ipotesi di creazione di un centro ad alta rotazione sull'altopiano carsico, di cui si è avuta notizia da un paio di giorni, si possa interpretare come un cambiamento radicale del Governo nella gestione degli arrivi dalla rotta balcanica, con la ripresa dei trasferimenti regolari da Trieste e dal Friuli-Venezia Giulia; se si possa definire superata la decisione di aprire un grande *hotspot* sul territorio regionale, annunciato a metà gennaio

e stabile ripresa dei trasferimenti, al fine di assicurare piena tutela della dignità e dei diritti fondamentali delle persone in arrivo e superare definitivamente l'attuale situazione di criticità riscontrata nell'area del Silos di Trieste

prorogato al momento fino al prossimo giugno. Il ripristino dei controlli, di cui non va sottovalutato l'effetto deterrente del fenomeno migratorio illegale, ha consentito sino al 12 marzo scorso, di respingere in quella frontiera 1.352 migranti a fronte dei circa 40 migranti riammessi in Slovenia nell'analogo periodo dell'anno precedente. La forte pressione migratoria via terra che si registra in quel quadrante geografico provoca ricadute anche sulla gestione dell'accoglienza, in particolare nella Provincia di Trieste. Di conseguenza, da tempo è stata posta in essere una strategia volta ad effettuare trasferimenti sistematici dei migranti in altre Regioni, con l'obiettivo di alleggerire le presenze nelle strutture di accoglienza di quel territorio. Nel 2023 dal Friuli-Venezia Giulia sono stati effettuati complessivamente 2.433 trasferimenti, dei quali 1.788 dalla Provincia di Trieste. Quest'anno, sui 685 trasferimenti dalla Regione, 348 hanno riguardato la Provincia di Trieste. Proprio nella giornata di oggi è previsto un ulteriore trasferimento di 50 richiedenti asilo. Secondo quanto riferito dalla questura di Trieste, un considerevole numero di migranti, dopo il primo contatto con gli uffici di polizia, non si presenta più per la successiva formalizzazione della richiesta di protezione internazionale. L'elevato impatto della pressione migratoria può pertanto determinare criticità come quelle della struttura dell'ex Silos dove si rifugiano migranti non collocati nel sistema dell'accoglienza o in posizioni irregolari sul territorio nazionale. Al fine di individuare una soluzione concreta e definitiva in sinergia con la proprietà, il Comune, la locale azienda sanitaria, i Vigili del fuoco e l'autorità giudiziaria, la situazione dell'ex Silos è alla costante attenzione della prefettura di Trieste, che ha acquisito all'inizio di quest'anno la disponibilità della proprietà a interventi di messa in sicurezza in vista della compravendita della struttura programmata nel mese di giugno. In tale prospettiva, nella seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dell'11 marzo scorso, dopo un'ulteriore disamina della questione, è stata valutata da parte del sindaco di Trieste la possibilità di adottare un'ordinanza di sgombero, nonché di perfezionare la concessione alla prefettura del campo *scout* sito nella frazione di Prosecco al fine di attrezzare una struttura di accoglienza capace di assorbire l'impatto della presenza di migranti sul territorio.

ma bisogna considerare che Trieste non è più città di confine e, quindi, forse andrebbe ripensato il sito dei controlli di Schengen. Le oltre 200 persone che dimorano nel Silos a fianco della stazione ferroviaria di Trieste vivono tra topi, fango e in assenza di servizi igienici. In questi giorni migliaia di persone hanno firmato una petizione indirizzata al Presidente della Repubblica che sarà a Trieste a metà aprile. L'accoglienza immediata dei richiedenti asilo privi di mezzi è dovere delle amministrazioni pubbliche, tanto alla luce del diritto internazionale e del diritto europeo, quanto alla luce della legislazione italiana. Non vengono assicurate nel caso dei rifugiati, costretti a riparare tra le mura diroccate del Silos, né la tutela della dignità e dei diritti umani, né la tutela della sicurezza e della sanità pubblica. che hanno portato la situazione all'attenzione nazionale e non solo, documentano la vergognosa, completa assenza delle istituzioni contrapposta alla straordinaria generosità dei volontari che apportano assistenza a esseri umani come noi. Ha ragione il vescovo di Trieste, monsignor Trevisi, quando parla di persone,

umiliati e offesi come persone, come uomini. Non si dimentichi, Ministro, che, se viene a mancare l'umanità, significa che il nostro Paese, per come viene gestito, in assenza di valori etici nei quali identificarsi come cittadini, è destinato al declino totale.

Ministro Crosetto, nelle settimane scorse è emerso un quadro inquietante, sconvolgente, di dossieraggio, di accessi abusivi e illeciti ai sistemi di sicurezza delle banche dati nazionali.

perverso di certa stampa (certi organi di stampa) e pubblici ufficiali infedeli, che vogliono avere conoscenza di informazioni riservate su politici, imprenditori e cittadini. Ministro, come già in passato vi è stata un'altra vittima di dossieraggi illeciti, ovvero Matteo Renzi (pensiamo soltanto alle assoluzioni di questi giorni del papà di Matteo Renzi *(Applausi)*, Tiziano Renzi, e di Luca Lotti, a cui va la nostra solidarietà,

più. Se così stanno le cose, se quello è il numero degli accessi che davvero sono stati fatti, in gioco c'è la sicurezza dell'intero Paese. Signor Ministro, la la sua opinione, rispetto ad un rischio oggettivo, ad un pericolo per la sicurezza nazionale e anche delle forze militari, a causa di fenomeni di questo genere. Il secondo quesito che le pongo è se

che una vicenda così importante meriti di essere approfondita e verificata all'interno di una Commissione d'inchiesta, la quale si occupi solo di questo, senza nulla togliere a ciò che, ovviamente, per la sua parte, sta facendo la magistratura e

quello che il procuratore Cantone ha chiamato un «verminaio». Pertanto, la mia risposta, per quanto riguarda questa parte, è quella del cittadino che ha denunciato. Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nazionale, non penso che ci siano, dietro questa vicenda specifica, delle problematiche che possano riguardare la sicurezza nazionale, dal punto di vista militare e della difesa del Paese. Ci sono altri tipi di problematiche qua esco dal ruolo di Ministro della difesa - che secondo me vanno al di là di questa inchiesta. Sono moltissimi i casi di accessi alle banche dati, fatti non solo in questa quantità e non solo in ambienti così prestigiosi, per cui sono state condannate e sospese persone in giro per l'Italia, negli ultimi anni. Lì c'è una una vicenda che riguarda l'abuso nell'accesso che fanno alcune persone, che hanno il potere di farlo per difendere il Paese o per cercare giustizia. Questo può riguardare delle responsabilità personali, oppure può riguardare un sistema di potere. Quando gli accessi non sono uno, ma sono migliaia e servono a formare dei *dossier*, in ambienti dove non è neanche prevista alcuna attività di indagine, quando questi *dossier* non servono ad alcuna attività di indagine perché non è aperta alcuna indagine vengono forniti ad altre persone non so per quale utilizzo, allora il Parlamento (secondo me il massimo luogo dove la democrazia trova compimento) deve interrogarsi sulle regole in atto, sulle persone che di queste cose possono abusare, sulle persone che su queste cose possono avere interessi, su come queste cose possono influenzare la vita democratica e politica, indipendentemente dalle parti.

su quali sono le logiche, le persone, gli interessi e il calcolo che ci sono stati dietro. Mi auguro che questo percorso sarà fatto. Che sia fatto con il Copasir, con la Commissione antimafia o con una Commissione speciale, non sta al Governo e non sta a me dirlo. Ma vorrei che il Parlamento, proprio per la democrazia, non per chi ha denunciato, arrivasse a ridefinire i confini e a far riprendere fiducia in tutte le istituzioni ai cittadini in questo momento. Le persone che amministrano la giustizia, la polizia giudiziaria, le persone che hanno accesso alle banche dati: tutti noi veniamo coinvolti da una delegittimazione complessiva in cui sembra che lo scontro di potere autorizzi chiunque a fare qualunque cosa.

Signor Ministro, intanto vorrei dire che siamo con lei non solo quando ci difende e quando esercita bene il suo ruolo di Ministro della difesa, ma anche quando definisce bene qual è il rischio della democrazia e del nostro Paese intorno a queste vicende. Vorrei sottolineare alcune questioni. Il tema è il seguente: esiste un sistema dietro questa vicenda? Naturalmente nessuno può immaginare che, per l'accesso enorme ad informazioni di quelle banche dati, questa vicenda riguardi soltanto un pubblico ufficiale curioso della vita di cittadini, politici, imprenditori. Questa vicenda riguarda la diffusione di informazioni attraverso organi di stampa ed è stata definita mercato illegale delle SOS con il coinvolgimento di organi di Stato di Stato e di stampa. Questa è una vicenda che ha una gravità inaudita e deve comportare il massimo dell'approfondimento e della verifica da parte della politica, senza timori,

e quindi del ministro Crosetto, c'è la credibilità delle istituzioni. Faccio un appello, signor Ministro, anche riprendendo le sue parole: il Parlamento prenda in carico la vicenda e la approfondisca in tutte le sedi opportune, compresa una Commissione d'inchiesta. Solo dopo aver recuperato la credibilità delle istituzioni e la verità, avendo scoperto davvero quale sistema e quanto profondo è, avremo capito alcune vicende anche della politica italiana. Parlo, ad esempio, della vicenda che ha riguardato il mio *leader*, Matteo Renzi, e della gravità delle accuse che sono state rivolte; parlo dei *dossier* fatti nei suoi confronti e di quanto vicende del genere abbiano purtroppo contagiato un'opinione su di lui e sulla politica. Difendere le istituzioni, difendere Matteo Renzi, difendere lei, ministro Crosetto, significa dare un contributo alla buona politica e alla difesa della nostra democrazia.

Signor Presidente, nei giorni scorsi l'istituto indipendente SIPRI ha pubblicato un rapporto sulle fluttuazioni nel commercio globale delle armi dal 2019 al 2023, da cui si ricava un quadro estremamente preoccupante che vede il nostro Paese protagonista in un settore che genera morte e distruzione.

L'impennata delle esportazioni italiane appare indice di una precisa volontà politica. Dato ancora più allarmante sono le zone di destinazione della vendita di armi, tra cui il Medio Oriente: un'area incontrollabile, teatro di conflitti brutali, a cui l'Italia sta, di fatto, contribuendo. A titolo di esempio, vorrei sottolineare che il Paese che importa la quota maggiore di armi è il Qatar, al centro di accuse per i suoi legami con Hamas. Poco utili appaiono, in tal senso, le condanne ai brutali attacchi del 7 ottobre, quando si è complici del sostegno che alcuni Paesi forniscono all'organizzazione che li ha compiuti. Ulteriore elemento di condanna è la fornitura di armi allo Stato di Israele, Paese in guerra, in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 185 del 1990. In merito, alcuni esponenti del Governo hanno dichiarato che l'Italia aveva interrotto l'invio di "qualsiasi tipo di arma" dall'avvio del conflitto. Un'affermazione smentita dai dati pubblicati da ISTAT sulle statistiche del commercio estero: tra ottobre e novembre 2023 l'Italia avrebbe infatti esportato "armi e munizioni" verso Israele per un valore di 817.536 euro, di cui una quota oscurata: tale mancanza di trasparenza dimostra come si tratti di armi e munizioni ad uso militare, poiché l'istituto,

A pagare le conseguenze di questa drammatica situazione in Medio Oriente è il popolo palestinese, con 31.000 vittime, di cui 12.000 bambini. Contribuire a un conflitto che sta provocando un tale disastro umanitario è inaccettabile per il nostro Paese e per le sue istituzioni. In un contesto come quello attuale, che vede l'innesco di numerosi teatri di guerra, tra cui uno nel cuore dell'Europa, chiedo al signor Ministro se intende chiarire gli orientamenti politici del Governo circa la produzione e l'aumento nell'esportazione di armi, indicatore di un cambiamento profondo degli equilibri; nonché se non intenda impegnarsi ad accrescere il livello di trasparenza in materia, al fine di contribuire all'efficacia del potere di indirizzo e di controllo parlamentare, chiarendo *in primis* se l'Italia abbia fornito o stia fornendo armi allo Stato di Israele dopo il 7 ottobre 2023.

In merito ai singoli quesiti, rispetto a quello sulle esportazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, titolare della materia, ha già spiegato

Questo è un fatto che, più volte, il Ministero e il Ministro degli affari esteri hanno ribadito e che io stesso ho ribadito. Contrariamente a quanto asserito, in occasione delle recenti riunioni dei gruppi di lavoro sul trattato sul commercio delle armi di Ginevra, l'Italia, insieme a Belgio e Spagna, è stata menzionata come Paese che ha adottato una politica di sospensione tempestiva e incisiva di trasferimenti di armi verso Israele dopo il 7 ottobre. L'Italia è stata Le licenze di esportazione verso Israele autorizzate prima del 7 ottobre erano già state in gran parte utilizzate, mentre su quelle non ancora utilizzate, cioè quelle già autorizzate prima, l'Unità per le autorizzazioni dei e non riguardano materiali che possano essere impiegati con ricadute nei confronti della popolazione civile di Gaza. Invece di cercare di inventare sterili polemiche, sarebbe stato giusto riconoscere che la Difesa e il Ministero degli affari esteri si sono profusi in uno sforzo umanitario e di sostegno alla popolazione civile di Gaza che non ha eguali nei Paesi occidentali, dall'invio della nave Vulcano agli assetti aerei a quello che stiamo facendo anche in questi giorni. Tornando al quesito, sia la posizione comune dell'Unione europea n. 944 del 2008, sia il Trattato per il commercio delle armi prevedono che la decisione di autorizzare o meno un'esportazione sia assunta sulla base di una valutazione del rischio che i singoli materiali possono rappresentare ai fini del loro utilizzo per commettere violazioni dei diritti umani, crimini internazionali o colpire la popolazione civile. Anche quando il Trattato, nei casi più gravi, prevede esplicitamente il divieto di esportazione, questo è riferito agli specifici materiali oggetto dell'esportazione e non a valutazione o o a previsioni generali sulla condotta di uno Stato. Vorrei concludere ricordando che l'impegno del Governo a rendere più trasparente ed efficace la legge n. 185 è già attuale grazie a un disegno di legge approvato da questa Assemblea in prima lettura il 21 febbraio scorso. Tra le misure previste viene ripristinato in forma aggiornata il Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la difesa, al fine di garantire il coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche per l'applicazione della legge n. 185. Nella relazione che il Governo dovrà necessariamente trasmettere al Parlamento, dovrà espressamente indicare l'indirizzo politico alla base delle relazioni assunte in materia di esportazioni. La reintroduzione dei comitati interministeriali è, peraltro, in linea con gli indirizzi contenuti nella relazione conclusiva, approvata all'unanimità dalla Commissione difesa del Senato nel giugno 2021. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

Come lei ben sa, nella passata legislatura è stata approvata - finalmente, a parer mio - la legge che dà la possibilità anche ai militari di unirsi in associazioni sindacali. In precedenza, era prevista la rappresentanza militare, i famosi Cocer. Per chi ci guarda e non conosce il tema, ricordo che la rappresentanza fungeva da cerniera e raccordo tra il personale, il comando e l'amministrazione difesa. Ad oggi, nell'attesa di una piena operatività e dei regolamenti attuativi discendenti, risultano iscritte nell'apposito albo presso il suo Dicastero circa trenta associazioni sindacali; mi corregga se non ho numeri aggiornati. alcune di tali associazioni siano guidate da dirigenti sindacali che svolgono contemporaneamente anche il vecchio ruolo di rappresentante Cocer. La prima domanda è, quindi, signor Ministro, se secondo lei questo doppio ruolo è legittimo. In una circolare del suo Dicastero di qualche tempo fa in cui si citava questa circostanza non è stato - a parer mio - dissipato o chiarito questo dubbio. Per cui rivolgo la domanda in maniera diversa: Ministro, mi conferma che sia preclusa la possibilità di ricoprire contestualmente i due ruoli, rappresentante Cocer e dirigente sindacale? Se la risposta è affermativa, in base a quale disposto normativo lo afferma? Signor Ministro, ritiene una possibile causa di rigetto della domanda di iscrizione all'albo delle associazioni il fatto che la dirigenza sindacale rivesta questo doppio ruolo? In ultimo, signor ministro Crosetto, le chiedo se rappresentanti Cocer non in servizio a Roma per l'espletamento del loro mandato ricevano compensi forfettari giornalieri a carico dell'amministrazione della e se in tal caso non si vengano a creare delle sperequazioni sostanziali con le associazioni sindacali che, invece, non hanno rappresentanti Cocer tra i propri dirigenti. Sappiamo che siamo in un periodo transitorio, ma non per questo possiamo creare differenti possibilità di esercizio del mandato sindacale tra le associazioni.*(Applausi)*.

puntualizzando che l'esclusione del duplice ruolo negli organi di rappresentanza e in quelli direttivi di associazioni sindacali è a legislazione vigente congrua e ragionevole, considerata la natura non sindacale degli organi di rappresentanza, costituiti anzi in funzione integrativa delle determinazioni dell'amministrazione sulle questioni di interesse personale. Mantenerli distinti serve per evitare confusioni di ruoli e a preservare il ruolo dialettico delle associazioni sindacali. In base a tale considerazione, se tale preclusione sia confermata e sulla base di quale disposto normativo; se la stessa possa costituire motivo di rigetto dell'istanza di iscrizione all'albo; se i rappresentanti Cocer non in servizio a Roma per l'espletamento del mandato ricevono compensi forfettari. In specifico riferimento a questi quesiti rispondo che la preclusione non è stata confermata da disposizioni normative o da successive circolari, come l'interrogante sa perfettamente. Fu il Governo *pro tempore* che ritenne opportuno non intervenire in questo caso. Tra il personale direttivo di alcune associazioni iscritte all'albo ministeriale vi è la presenza di militari eletti nella rappresentanza militare, e glielo confermo. Così i rappresentanti Cocer, quando svolgono il mandato rappresentativo al di fuori della propria sede di servizio, al pari di qualsiasi militare comandato in servizio isolato, hanno diritto al rimborso delle spese di missione. ricorrendone i presupposti, hanno facoltà di richiedere all'amministrazione di appartenenza la corresponsione di una somma forfettaria, a titolo di rimborso ai sensi articolo 7, comma 9, In merito all'asserita sperequazione che l'interrogante evidenziava, io ribadisco che non questo Governo, ma quello *pro tempore* ritenne opportuno non intervenire e rimandare all'eventuale intervento legislativo il compito di superare tale condizione, che non c'è stato né prima né dopo. Il Governo prende atto di questo e non può da parte sua dare interpretazioni che superino la legislazione. Segnalo infine - questa è la notizia positiva - che è in corso il procedimento di accertamento delle organizzazioni sindacali rappresentative, a seguito del quale cesseranno le funzioni della rappresentanza militare, in un continuo per cui non si sovrapporranno mai l'una all'altra. Ed è probabilmente il motivo

Signor Ministro, prendo atto della sua risposta. Nella stesura della legge sulle associazioni sindacali, io avrei fatto altro tipo di scelte e posso immaginare che probabilmente anche lei avrebbe fatto altre scelte. Il risultato - a mio avviso - è stato un compromesso. Non è una sua responsabilità. però, Ministro, visto che è lei in questo momento a fare gli attuativi, che questi vadano nella direzione di piena ed effettiva operatività dei diritti sindacali, seppur nella specificità che il mondo militare rappresenta. Magari in un futuro prossimo, in altra occasione, sempre in ottica di tutela piena ed effettiva del personale, ci confronteremo anche sulla previdenza dedicata e sul sistema di avanzamento delle carriere di tutto il personale della Difesa, militare e civile. In ultimo, per cortesia istituzionale, le preannuncio un'interrogazione che spero attiverà gli uffici per una pronta risposta relativamente alla qualità delle acque nelle nostre navi militari. Parlo delle acque ad uso umano per il personale imbarcato.

del ministro Crosetto,